Ieri il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che dobbiamo smetterla di guardare bozze e documenti non ufficiali per commentare il disegno di legge di bilancio. Questo è il Senato della Repubblica e avrebbe dovuto ricevere

non sa oggi - e deve commentare documenti non ufficiali e bozze - perché la legge di bilancio è sparita. Allora chiedo al Ministro per i rapporti con il Parlamento - perché questo incide sull'ordine dei lavori di quest'Assemblea per le quando tornerete in Consiglio dei ministri per approvare il testo definitivo. Se quelle sono bozze e quest'Assemblea non ha ancora ricevuto nulla, vuol dire che o quel documento è stato approvato salvo intese e quindi torna in Consiglio dei ministri, oppure è stato approvato definitivamente e quindi ci chiediamo come mai dopo undici giorni non è arrivato al Senato della Repubblica, che deve discuterlo.

così come è stato sottovalutato l'intero sistema della devianza criminale giovanile, che non ha confini. Mi soffermo su un dato: dalla fine del 2022 i numeri dei giovani reclusi nelle nostre carceri minorili sono spaventosamente aumentati e sono aumentati i casi di *baby gang*,

che è nata per l'indifferenza dello Stato e che ha creato indifferenza alla prepotenza. Quindi, abbiamo deciso di intervenire su Caivano, dove c'era un allarme, ma intendiamo farlo con questo provvedimento anche sull'intero Paese, per evitare altre Caivano. di decidere, abbiamo finalmente e doverosamente deciso di intervenire per riportare di moda le regole ed il rispetto, ma l'abbiamo fatto consapevolmente intervenendo su due direttrici: una, quella importante che molti di voi hanno ricordato, è la prevenzione. L'abbiamo fatto in questo provvedimento faccio specifico riferimento ad alcuni strumenti che abbiamo introdotto per la devianza e la criminalità giovanile. Vi è l'ammonimento, che è uno dei primi provvedimenti che abbiamo voluto adottare, con un'incidenza non tanto e non solo nei confronti dei giovani, anche dodicenni, quindi dai dodici ai quattordici anni, ma soprattutto per coinvolgere i genitori; l'abbiamo fatto con il Daspo, l'abbiamo fatto con l'avviso orale, l'abbiamo fatto

L'abbiamo voluto anticipare per potenziarlo e poterlo applicare prima. Abbiamo voluto operare anche interventi sul lato della repressione, certo, ma con strumenti di buon senso contro i fenomeni di spaccio, anche di lieve entità, contro i fenomeni odiosissimi di *stesa* che accadono proprio in certi territori, contro una messa alla prova che non funziona quando siamo in presenza di reati gravissimi (stiamo parlando di omicidio pluriaggravato, di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata, di rapina pluriaggravata). nei confronti del fenomeno dell'abbandono scolastico, ma ancor di più siamo intervenuti sul sistema carcerario o di esecuzione penale minorile abbiamo deciso di farlo, tirandoci su le maniche, avendo il coraggio di dire che le cose non vanno

Parlo di strutture di IPM - lo dico io che ho la delega su questo tema

che devono essere adeguate a fare vera educazione, perché non stiamo parlando di rieducazione, bensì di strutture capaci di fare vera educazione. Questa educazione, della quale tutti parlano, non si può fare all'interno delle carceri che noi abbiamo ereditato e dalle quali escono i ragazzi in fuga. Vi ricordate il Beccaria a dicembre dell'anno scorso? Ci

Treviso e investire in un progetto unico nel suo genere che sarà quello dell'IPM di Rovigo, che non sarà un carcere come quelli che abbiamo ereditato dal passato, ma sarà una struttura capace di fare vera educazione, attività, formazione e lavoro. A questo ci siamo dedicati. La soluzione non sta ovviamente nel far finta di nulla, non sta nella visione che non c'è, ma dobbiamo leggere i numeri e individuare delle soluzioni, trovando il coraggio anche di avere una visione di insieme, perché la giustizia arriva quando ormai il danno è stato fatto. Dobbiamo lavorare insieme pensando che l'educazione minorile è una risorsa di questo Paese ed è una risorsa per tutti noi, quindi la giustizia deve lavorare con la scuola

anche coinvolgere i genitori in questa operazione. Riportiamo al centro le regole e il rispetto, temi che noi intendiamo ovviamente riportare di moda, ma intendiamo farlo anche con il contributo di chi, anche dalle opposizioni, vuole e ha voluto dare una mano. Per questo prima ho detto che i ringraziamenti li faccio alla fine. Ringrazio le opposizioni perché in questo lavoro, che abbiamo fatto insieme, dalle opposizioni sono arrivati dei suggerimenti che abbiamo accolto, certo non tutti, ma dei suggerimenti sono arrivati e alcuni sono stati accolti, così come sono stati accolti i suggerimenti che sono arrivati grazie alle audizioni che abbiamo svolto. L'articolo 27-*bis* sulla messa alla prova anticipata l'abbiamo migliorato, ma l'abbiamo fatto insieme e credo che questo sia il giusto modo di operare, perché il Parlamento, in questo caso specifico, non è stato esautorato, ma ha partecipato.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, nel testo proposto dalle Commissioni riunite

Manteniamo un livello civile del dibattito.

-, ma questa legislatura ha già superato le tre legislature precedenti. Siccome le tre legislature precedenti erano state caratterizzate da storie di tutti i tipi, chiedetevi che cosa succede dentro questa maggioranza. Chiedetevi su cosa non andate d'accordo. *(Applausi)*. Signor Presidente, il decreto-legge bandiera della presidente Meloni ed è finito male, peggio di tutti gli altri, con una richiesta di fiducia che non è posta sulle richieste dell'opposizione, visto che il sottosegretario Ostellari,

messa contro la stessa maggioranza. *(Applausi)*. È evidente che soprattutto Lega e Fratelli d'Italia parlano lingue diverse. È evidente che ci sono fratture che sono sotto gli occhi di tutti. Signor ministro Ciriani, apprezziamo la sua consueta disponibilità e dedizione all'attività quotidiana del Parlamento, ma se siamo a 34 fiducie poste, tre al mese,

e temo - lo anticipo, presidente Centinaio - che la settimana prossima dovrà essere dedicata ad una valutazione profonda e seria su come intendiamo andare avanti. La legge di bilancio infatti in queste condizioni non può essere affrontata; lo diciamo prima per evitare di essere tacciati poi per coloro che fanno ostruzionismo o resistenza perché non la facciamo, vogliamo entrare nel merito, vogliamo discutere. Come ha detto però il presidente Patuanelli prima di me, sono passati giorni e la conferenza stampa della presidente Meloni è stata completamente cancellata dai provvedimenti. La prego, signor Presidente, di far presente al presidente La Russa che se non otteniamo i testi in queste ore, saremo obbligati ad iniziare audizioni informali fuori dal Palazzo con chi non conosce ancora i tratti di questa manovra. Lo abbiamo detto più volte. Non diteci la prossima settimana che siamo eversivi o non siamo in linea con le regole del Parlamento perché saremo obbligati a iniziare le audizioni in maniera informale e autonoma. Signor Presidente, la prego di far presente al presidente La Russa che noi pretendiamo i testi della manovra e le relazioni tecniche in queste ore perché siamo stanchi di sentire le cose che dice il vicepremier Salvini, salvo poi essere smentito dagli uomini e le donne che fanno capo alla Presidente del Consiglio. Va avanti così da un anno. Non è più accettabile.

nel testo proposto dalle Commissioni riunite 1a e 2a. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato più di un mese dal primo *blitz* compiuto dalle Forze dell'ordine nel Parco Verde di Caivano, a cui ne sono seguiti altri. Sono state effettuate decine di perquisizioni, al termine delle quali sono state sequestrate cocaina, *hashish*, armi e munizioni, denaro contante, impianti di videosorveglianza con telecamere poste a vigilanza di locali ed aree esterne. La presenza della presidente Meloni nel Comune campano ha indubbiamente smosso le acque su una condizione di degrado che si protraeva da anni e sulla quale non era più procrastinabile il dovere di intervenire. Non si trattò solo di una passerella, perché a seguito di quella visita sono stati compiuti i fatti, e non solo con i *blitz* delle Forze dell'ordine, ma anche con l'arrivo di insegnanti e funzionari comunali e ovviamente con il rafforzamento dei presidi di sicurezza. Con questo decreto il Governo ha inteso dare una risposta forte dopo l'avvenuto stupro ai danni di due giovanissime ragazze, introducendo misure cautelari per minori, Daspo urbano, foglio di via, misure di contrasto alle *baby gang*, ammonimento, misure sul processo penale a carico di imputati minorenni e istituti penali per minorenni. Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle *baby gang*, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'avviso orale. Attualmente la misura è prevista per i soggetti maggiorenni, che per la condotta e il tenore di vita si ritiene vivano anche in parte con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme l'avviso orale si è reso applicabile anche ai minorenni, a partire dai Si prevede che il questore possa proporre all'autorità giudiziaria di vietare a determinati soggetti di età superiore ai quattordici anni di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce, quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni, maggiorenni, il tutto al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento. Si rafforza l'offerta educativa nelle scuole del Meridione, caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggior disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione di quelli che permangono nella stessa istituzione scolastica, garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti, quali l'attribuzione di una quota pari al 50 per cento dell'incremento del fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica, e l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di dieci punti a conclusione del triennio effettivamente svolto e ulteriori due punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio. Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento e dell'obbligo scolastico. Si introduce una nuova fattispecie di reati per i casi di elusione; nell'ipotesi di dispersione assoluta, si introduce la pena fino a due anni di reclusione; in caso di abbandono scolastico, la pena prevista è fino a un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione. Quelli che ho elencato sono solo alcuni dei provvedimenti contenuti in questo decreto-legge, nel quale il Governo ha proceduto su un doppio binario: avanti a tappe forzate sul progetto di riqualificazione del centro sportivo Delphinia, il luogo degradato a ridosso del Parco Verde in cui si sono consumate orribili violenze ai danni di due cuginette; in contemporanea, però, avanti anche sulla stretta penale per i minori che delinquono, tra gli altri, il reato di *stesa*, che consiste in un corteo di giovani che a bordo di motociclette attraversano i quartieri a forte velocità, esplodendo in aria colpi di armi da fuoco per dimostrare la propria forza sul territorio e lanciare un messaggio di impunità. Finora la *stesa* era un'aggravante rispetto ad altri reati, ora immaginiamo di trasformarla in un delitto autonomo. Caivano vuole rappresentare un esempio di come lo Stato intende contrastare ovunque la presenza territoriale del crimine organizzato. Questo decreto-legge costituisce solo un primo passo verso quella che per noi costituisce una vera e propria missione per ridare soprattutto al Sud una dignità sociale spesso compromessa a causa delle mafie.

vigili urbani, vinse il bando per la riqualificazione delle periferie dei fondi nazionali Pinqua, entrando in graduatoria. I soldi, però, ahimè, sono finiti prima e il progetto non è mai partito. Opportunità di lavoro inesistenti, stabili fatiscenti, la classica situazione, purtroppo, di molte periferie del Sud. Vede, Presidente, a dispetto di quanto racconta la propaganda governativa, questa lettera, di cui ho citato qualche passaggio, è immediatamente successiva alla cerimonia del passaggio della campanella tra il presidente Mario Draghi e la nuova presidente Giorgia Meloni. La lettera, come si vede dal protocollo, è datata 24 ottobre 2022, cioè esattamente un anno fa. Signor Presidente, a questa lettera la presidente Meloni rispose promettendo una visita, ma questa promessa non fu mantenuta, perlomeno fino agli ultimi drammatici fatti, che hanno poi ovviamente scosso le coscienze di tutti e hanno determinato la successiva visita. Come si vede, al di là della retorica e delle bugie che sono state raccontate nelle ultime settimane, quando serviva il Governo a Caivano non c'è andato. Ha aspettato che succedesse l'ennesima tragedia prima di fare quella che è somigliata davvero a una passerella, una operazione di propaganda a colpi di *spot*, come peraltro è successo molte volte in questo primo anno di vita del Governo: l'ennesima tragedia, l'ennesima passerella e anche l'ennesimo decreto-legge. In questo caso, peraltro, come è stato osservato tante volte in Commissione, il decreto-legge è ancora più discutibile dal punto di vista dello spirito costituzionale, come tutti quei provvedimenti che riguardano le libertà personali, personali, che dovrebbero essere rigorosamente approvati con legge ordinaria e non attraverso la decretazione d'urgenza, di cui invece questo Governo sta abusando a piene mani, come mai prima d'ora nella storia della Repubblica, peraltro ponendo sempre la fiducia, come ha fatto questa mattina. Ma di questo abbiamo già discusso nella giornata di ieri, quando abbiamo avanzato la questione pregiudiziale di costituzionalità, quindi non aggiungerò altre parole. Voglio, invece, affrontare un punto più di merito e, in particolare, contrastare, almeno dal mio punto di vista, la concezione totalmente sbagliata che attraversa questo provvedimento, ossia l'idea che, all'indomani di fatti di cronaca di particolare disvalore e di particolare allarme sociale, si coltivi l'illusione di inseguire questa o quella emergenza attraverso l'irrigidimento degli strumenti penali. Insomma, il carcere come soluzione a tutti i problemi, anche se, come sappiamo, la storia di questi anni ha dimostrato come l'aumento delle pene non sia la soluzione più efficace per contrastare i fenomeni criminali. Signor Presidente, io che pure sono cresciuto e ancora mi riconosco totalmente in quella bellissima frase, che abbiamo ascoltato più volte in questi giorni, secondo la quale, prima di ogni altra cosa, servirebbe l'esercito di assistenti sociali, di psicologi, di maestri di strada, non credo affatto che non servano anche gli strumenti più tipici dell'azione penale o che non si debba far sentire la presenza dello Stato. Certo che servono: serve la legge, servono i magistrati, servono le Forze dell'ordine; nessuno lo ha mai negato e nessuno ovviamente potrebbe mai negarlo. Ma lo Stato non può essere soltanto repressione. *(Applausi)*. Lo Stato è anche la scuola, il lavoro, il tempo pieno, gli spazi sociali, lo sport, gli asili nido, le mense, le biblioteche. Serve allora soprattutto un equilibrio,

sceglie un approccio totalmente securitario, introduce norme penali che, peraltro, come è evidente che sia, riguardano non solo Caivano ma tutto il territorio nazionale, utilizza la sanzione penale come prima e sostanzialmente unica risposta al disagio sociale e al disagio minorile, pretendendo che il timore di una condanna funzioni come un deterrente rispetto a condotte di adulti e di minori che sono, però, espressione di una privazione profondissima. Tale privazione ha radici anche nelle condizioni di vita, nella povertà sociale, culturale ed educativa di un contesto sociale che spesso è disperato, degradato e segnato anche da una diseguaglianza strutturale - mi rivolgo al Governo, con un inciso - il vostro scellerato progetto di legge sull'autonomia differenziata ovviamente accentuerà. Eppure, chi conosce i minori che vivono nei contesti di disagio ci ha detto chiaramente che la strada della repressione, dell'innalzamento delle pene edittali, spesso o almeno quasi sempre, si rivela del tutto inefficace, soprattutto quando la trasgressione delle regole è, nei percorsi di vita, un preciso modo di essere, che il più delle volte ribadisce l'appartenenza ad un sistema ambientale o ad un sistema familiare che, per certi versi, purtroppo sopperisce anche all'assenza delle istituzioni. Il decreto interviene sulle famiglie solo sanzionandole e, da questo punto di vista, una vera e profonda incoerenza tra le misure adottate in caso di mancato assolvimento dell'obbligo scolastico e l'assenza di qualsiasi misura di supporto o di intervento formativo e sociale rispetto alle famiglie. Per l'appunto, la sola circostanza che questo gravissimo fatto accaduto a Caivano, un caso di violenza contro le donne, anzi contro donne giovanissime, non preveda immediatamente misure più specificatamente volte a contrastare la violenza di genere, mi pare, anche questo, molto indicativo. Non si cita mai, nemmeno come riferimento, l'educazione di genere, che pure è un tema chiave o dovrebbe essere un tema chiave per intervenire in una prospettiva di prevenzione e di contrasto al disagio giovanile e alla violenza. *(Applausi)*. Non sono previste misure volte all'educazione alla cittadinanza.

una porcheria contro cui fare muro l'educazione sessuale nelle scuole. È stato detto ieri, in un delirio oscurantista, e perciò davvero non ci si meraviglia più di tanto. Insomma, nella filosofia di questo decreto-legge c'è veramente un'idea di Paese, la vostra idea di Paese, che, dal mio punto di vista, è completamente sbagliata: un Paese in cui debbano prevalere soltanto risposte punitive e repressive, non quelle educative e preventive. Gli investimenti in risorse culturali, come quelle incentivanti per gli insegnanti, tanto per citare una questione seria, benché menzionati nel provvedimento, hanno l'enorme limite di essere concepiti soltanto come misure emergenziali e non strutturali. Le misure sanzionatorie, invece, il risultato che si avrà l'effetto di aggravare la situazione delle strutture carcerarie minorili che pure, come sappiamo, dovrebbero essere, in particolare nella giustizia minorile, una vera e propria *extrema ratio*. Ciò è in aperto contrasto con quello che è un principio fondamentale del sistema penale, principio che impone peraltro una indagine accurata sulla personalità del minorenne, per evitare i cosiddetti effetti stigmatizzanti della condanna al carcere, e che impone la predilezione delle misure alternative. Pensiamo, per esempio, all'istituto della messa alla prova; istituto, peraltro, che in un tempo nemmeno particolarmente lontano, alcuni anni fa, si immaginò di estendere alla giustizia degli adulti e che invece oggi viene radicalmente messo in discussione anche per i minori. Quindi, davvero è un'inversione di tendenza clamorosa. Una idea di sicurezza, dunque, che ruota solo attorno all'idea della punizione e della repressione. Una idea che interviene anche aumentando la pena minima da sei a diciotto mesi per i fatti di lieve entità in tema di stupefacenti, in particolare Certamente io non mi aspetto da voi quello che ormai si sperimenta in molte parti del mondo, cioè la legalizzazione delle droghe leggere, che, dal mio punto di vista, è l'unica vera forma di contrasto alla criminalità organizzata.

probabilmente meno oscurantiste delle destre italiane, o comunque forze politiche non certamente ascrivibili al campo progressista. Per tutte queste ragioni, di metodo di merito, per la scelta di non puntare minimamente sugli aspetti che dovrebbero essere, quelli sì, sì, davvero centrali e decisivi, io annuncio il convinto e totale dissenso su questo provvedimento da parte del mio Gruppo e quindi il voto contrario dell'Alleanza Verdi

sta soltanto ratificando norme. Devo dire che questa volta siamo stati anche la Camera - per così dire - fortunata, perché oggi è il 27 ottobre; questo provvedimento arriverà alla Camera il 6 novembre e scadrà il 15 novembre, quindi rivolgo un saluto affettuoso ai colleghi deputati che dovranno semplicemente mettere un timbro sul nostro lavoro. Però una volta capita a loro e una volta capita a noi: sappiamo di vivere in un regime di bicameralismo del tutto fittizio, quindi va così.

un modo di manifestare l'identità stessa di questo Governo. Il metodo adottato nell'assunzione di questo provvedimento è proprio il modo in cui il Governo lavora. Quindi credo che il nostro voto su questo provvedimento in realtà in realtà vada a toccare certo il merito del provvedimento, ma anche un modo di fare, un modo di vedere questo Paese. Questo è un provvedimento che nasce da un evento di cronaca terribile, che ha colpito naturalmente le emozioni di tutto il Paese: la violenza contro due ragazzine, la violenza la violenza portata contro queste due giovanissime da un gruppo a loro volta di giovanissimi. Si tratta di un evento di cronaca terribile che però significava anche un grido di allarme, in un certo senso, poiché era il segno che in certe nostre periferie esiste una situazione di degrado, di marginalità e di devianza che è davvero arrivata a prefigurare scenari che descrivere fa gelare il sangue nelle vene. Quale sarebbe stato, secondo me, l'atteggiamento di una classe dirigente responsabile? Sarebbe stato quello di assumere questo problema, analizzarlo a fondo, reperire dati, discutere le cause di tutto questo e mettere in campo una proposta per tutte le periferie del Paese che avesse un senso di crescita e di sviluppo; che andasse a guardare alle cause e alle radici del problema; che rimuovesse insomma non soltanto il sintomo di quella marginalità, di quella povertà, di quell'assenza di lavoro che provocano poi quegli eventi di cronaca, ma anche le cause di quegli eventi di cronaca e quindi risolvesse quella marginalità, quella povertà educativa, quell'assenza di lavoro. Invece il Governo cosa fa? Quello che fa di solito. va sul posto - naturalmente la Presidente del Consiglio, con tutta la sua buona fede, non ha potuto incontrare neanche uno degli abitanti di Caivano perché, quando la Presidente del Consiglio va in un posto del genere, il cordone di sicurezza è tale che l'interazione è minima - e, come era già successo a Cutro e anche

Qualcuno dai banchi della maggioranza ha detto: abbiamo ritenuto che fosse il caso di agire d'urgenza. Ma ai colleghi della maggioranza dico che la Costituzione non è che si applica quando si ritiene; la Costituzione si applica se l'urgenza c'è, non quando si ritiene di doverla applicare perché secondo qualcuno c'è l'urgenza. Allora si sarebbe dovuto avere un provvedimento pensato, ma questo è tutto il contrario di un provvedimento pensato. È un provvedimento che purtroppo è soltanto una forma di propaganda, forma di propaganda, perché si occupa soltanto di un Comune, solo del Comune di Caivano. Ne ha bisogno il Comune di Caivano? Certamente. Va benissimo poter intervenire a favore del Comune di Caivano, ma abbiamo risolto il problema delle periferie, abbiamo risolto il problema di tutti i Comuni che sono accanto al Comune di Caivano e che vivono situazioni ugualmente complicate? Quando un decreto del Governo decide di dare nuovo personale e nuove risorse al Comune di Caivano, cosa diciamo ai Comuni accanto? Cosa diciamo alle mille periferie di tutto il Paese? Cosa diciamo alle periferie della capitale? Cosa diciamo alle periferie anche delle zone più prospere prospere del Paese? Ci sono Caivano in tutta Italia. Ci saremmo aspettati un'analisi e un piano organico, come quello che fu varato nel 2016, il piano periferie d'Italia, pensato dal nostro collega Renzo Piano, ispirato dalla sua azione: il piano che mise a disposizione 2 miliardi per interventi per le periferie, creando strutture che ancora oggi insistono sui nostri territori e che sono andate lì direttamente a risolvere il problema; un piano che sciaguratamente è stato messo via. Sarebbe stato importante che questo Governo, un Governo politico - ci viene detto avesse pensato in modo strategico. Invece si va a Caivano, si dice quindici vigili urbani, dopodiché misteriosamente in Commissione si ritira, per esempio, un emendamento dei relatori che prevedeva 10 milioni di di incentivazioni e di esenzioni fiscali e contributive per gli imprenditori e i professionisti di Caivano: un emendamento scritto sull'acqua che non è mai stato approvato. Quindi, le risorse sono state anche molto minori di quelle che si pensava e si immagina di aver risolto il problema, insistendo su un singolo Comune in un'area estremamente complicata. Ma il Comune è soltanto quello e questa è una gamba del decreto, quella che avrebbe dovuto essere la promozione. C'è una seconda gamba del decreto, che non si occupa soltanto di Caivano: è quella parte che si occupa di giustizia minorile. Perché se i minori di Caivano vengono sostenuti e poi puniti, i minori di tutto il resto del Paese vengono soltanto puniti,

senza il ragionamento che anche il lavoro sulla libertà dei cittadini dovrebbe richiedere, la serietà della riflessione che si dovrebbe fare quando si incide sullo stato di libertà dei cittadini. Che cosa si fa? Si prendono i nostri ragazzi, che, per quanto

sulla loro educazione. Quando pochi minuti fa il Sottosegretario è intervenuto e ha detto che hanno pensato alla prevenzione, la prevenzione per voi è il Daspo, la prevenzione è l'ammonimento.

di una marginalità gravissima, dell'assenza delle famiglie e della loro incapacità, anche per mancanza di mezzi, di seguire quell'educazione. La prevenzione sta nel rimuovere le cause del crimine e della devianza, non soltanto nel punire il crimine e la devianza. Che cosa c'è in questo Avete deciso, al contrario di quello che si era fatto sinora cioè utilizzare i migliori istituti della giustizia minorile per estenderli alla giustizia degli adulti, di fare il contrario ed equiparare sempre di più ragazzi

Li porteremo nelle prigioni minorili. Abbiamo sentito il garante per i detenuti, Mauro Palma, dirci che ci sono 428 posti negli istituti penali per minori e 427 occupati. Questa è la visione di una risoluzione semplicistica di problemi gravissimi, una visione che non andrà ad attaccare i problemi del Paese: i problemi sociali, i problemi economici e anche i

che esiste a Caivano, esiste nei paesi vicini e che resterà identica, salvo aver dato l'occasione a qualcuno di fare delle fotografie e mostrarsi ai cronisti.

rappresentanti del Governo, colleghi, vedete, c'è un limite anche alla polemica e alle bugie che stiamo ascoltando. Prima considerazione: chiedete perché si mette la fiducia. Ieri ho seguito sia nel ruolo di Vice Presidente, sia come rappresentante, insieme ai miei colleghi, del Gruppo Forza Italia, l'andamento dei lavori e avendo avuto una lunga discussione in Commissione che ha anche visto l'attenzione - doverosa - alle motivazioni e alle proposte delle minoranze,

un cortese assistente, una copia del provvedimento): nel testo si parla di scuola, di istruzione, di legalità, di famiglie, non solo di punizione. E allora non venite qui a dire bugie. Il Governo interviene più sulle scuole che sui commissariati di Polizia, quello che voi non fate, quello che voi non sapete. Leggetevi il provvedimento. Siete talmente impegnati ad abbaiare che non avete tempo di leggere. Questa è la verità.

Ho già ripreso il presidente Gasparri sull'affermazione e ha annuito. Di conseguenza, per me la situazione è già ripristinata. Per favore,

in questo provvedimento ci sono interventi per le scuole e c'è il richiamo ai genitori, perché un genitore che sottrae il figlio alla scuola va punito severamente, non va incoraggiato come vorreste voi. Questo c'è scritto nel testo. Qualcun altro ha parlato di passerelle. Bugiardi (si può dire?)! Il Governo non è andato solo a fare la conferenza stampa, io leggo tutti i giorni del sottosegretario Mantovano, del ministro Bernini, del ministro Piantedosi, del ministro Valditara che vanno lì a dare attuazione alle norme del decreto-legge, questa è la verità. *(Applausi)*. Non sono le vostre passerelle, è l'azione di Governo su scuola, università, commissariati. Serve lo sport, andate a vedere le immagini delle ruspe delle Forze armate che hanno iniziato la demolizione e la ricostruzione di un centro sportivo. C'è un limite alla menzogna, anche nel Parlamento. Questa è la verità.

cari amici e colleghi. *(Applausi)*. Questo è un provvedimento di ampio respiro, che basta leggere per vedere quanto e come si occupa di scuola, istruzione, sport, lotta alla droga. Ma chi governava a Caivano? Chi è il Presidente della Regione Campania? Chi è? Non è governata? È del vostro partito, dissidente, ma viene dal PD. E, allora, scusatevi per l'inerzia del PD e di De Luca che nulla hanno fatto per l'emergenza Caivano, *(Applausi)*. Potremmo parlare anche di Gualtieri, che ha fatto il sindaco controvoglia e dovrebbe occuparsi di altre periferie, Tor Bella Monaca e altrove, dove questo Governo sta rafforzando la presenza dello Stato. Voglio anche ringraziare

ci sono stati e ci sono i don Patriciello e i don Coluccia che fanno quello che i De Luca e i Gualtieri non fanno sul territorio. *(Applausi)*. Grazie don Patriciello. Grazie don Coluccia. Invece don Vincenzo sta a Salerno o non so dove; mi riferisco a De Luca. È intento forse a designare parenti in giunte e Parlamenti.

Noi siamo quelli del recupero e della prevenzione. Noi siamo quelli che stanno dalla parte delle comunità terapeutiche che danno la vita; voi, invece, vorreste legalizzare le droghe. Ora in Campania c'è il procuratore della Repubblica Gratteri, andate a sentire le sue conferenze, dove vi spiegherà che la legalizzazione delle droghe non scalfisce gli affari delle cosche, ma li alimenta. Andate a sentire Gratteri se non volete sentire noi e imparate la verità. Il provvedimento verità. Il provvedimento è ricco di spunti e di impegno. Il Governo non fa passerelle perché va tutti i giorni a fare quello che questo decreto-legge impegna a fare. La questione non riguarda solo Caivano; le periferie con problemi sono tante e numerose. Nella città di Roma, da dove parliamo, ce ne sono tante. Ci sono in tante parti d'Italia, anche al Nord perché non è un problema solo del Sud. è inoltre un problema solo di repressione. La malafede, cari colleghi, ha un limite. Capisco che non avete letto il provvedimento, ma leggetelo perché si parla di scuola, d'istruzione, di obbligo scolastico. Ci sono interventi sullo sport, sulla salute, sugli psicologi, su quello che serve. Sappiamo bene infatti che non basta solo la repressione. Dopodiché se il provvedimento non piace a Saviano, ce ne faremo una ragione. *(Applausi)*. Ha detto che va via dall'Italia e resteremo in numero sufficiente per mandare avanti questo Paese. Ne leggo tanti, di questi partenti che restano in Italia; appena vince il centrodestra c'è un elenco di annunci e partenze. partenze. C'era Berlusconi, vado via; c'è la Meloni, vado via ancora prima. Poi restano tutti qua e noi siamo contenti *(Applausi)*; restino qua perché questo Paese è governato meglio e converrà anche a loro stare in Italia. Se poi vogliono andare via, ognuno è libero di farlo. Si muovono tutti: clandestini, turisti, italiani, stranieri; chi vuol viaggiare, viaggi, chi vuole restare, resti. Mi auguro che restino, perché è bene stare in Italia. L'Italia è un gran bel Paese. Cari colleghi,

Presidente, i richiami valgono solo per me o anche per loro? Io sono esperto di Aula, quindi non mi spavento. Ci attendiamo delle proposte e delle puntate di «Report». In questa legislatura, colleghi, si fanno operazioni trasparenza. Si stanno facendo in Commissione antimafia su alcuni magistrati che archiviavano parte delle inchieste di Borsellino le facciamo su Caivano e sulla lotta alla droga. È una legislatura della verità, della trasparenza e della legalità, cari colleghi! Fate quindi quello che giustamente ritenete di fare. A me non scandalizza nemmeno l'ostruzionismo, è normale fare 340 o 3.400 emendamenti, l'ho fatto anche io. C'è poi il Regolamento, con la fiducia e la necessità di discutere. Anche io sono dispiaciuto del fatto che i decreti-legge abbiano un esame monocamerale.

con una presenza adeguata del Governo: io sono quindi per la centralità del Parlamento, ma anche per la centralità della verità. Forza Italia con orgoglio voterà a favore del provvedimento in esame e ringrazio i colleghi del nostro Gruppo, il relatore e tutti quelli che hanno contribuito a renderlo migliore. Sappiamo di non aver risolto un'emergenza, ma di averla affrontata; addirittura qualcuno diceva che non bisognava fare il provvedimento contro i ragazzi che vanno in giro, aizzati dalla camorra, a sparare con i mitra, a fare la cosiddetta *stesa*. Qualcuno vuole la droga legale e la stesa tollerata. Noi siamo per la legge, l'ordine, l'educazione, la scuola, l'obbligo scolastico, la salute, lo sport e il coraggio che lo Stato deve avere, *(Applausi)*, perché non possiamo delegare solo a figure religiose. Ricordo padre Rastrelli, un altro sacerdote che lottava contro l'usura

Ne ha facoltà, ricordando ai colleghi che ci si rivolge sempre alla Presidenza. Mi scuso con il senatore Gasparri se prima non ho interrotto i colleghi, ma la questione dei partenti mi ha fatto ridere e me ne scuso. Signor Presidente, proprio a lei volevo rivolgermi per condividere con lei, che sono certa mi comprenderà, la difficoltà che provo in questo momento a dover parlare di un tema così delicato, così doloroso, così profondamente sentito (ne è dimostrazione il grande lavoro che è stato fatto fino a notte tarda nelle Commissioni riunite su questo provvedimento) dopo

ha dato a noi degli spacciatori, dicendo che diamo la droga ai ragazzi. *(Applausi)*. Io ho serie difficoltà a parlare dopo il presidente Gasparri, che si è detto esperto d'Aula, ma in realtà è esperto di insulti, sapendo di poterla passare liscia perché ha l'immunità parlamentare. *(Applausi)*. Attraverso di lei, signor Presidente, mi permetto allora di consigliare, come ha fatto il nostro senatore Scarpinato, al presidente Gasparri di rinunciare all'immunità parlamentare e poi vediamo se continua a essere così esperto di insulti.

solo da una settimana nelle Commissioni, perché questi purtroppo sono i tempi previsti dalle conversioni dei decreti-legge. Sono tempi molto ristretti. alcuni di noi, quelli che hanno la ventura di essere nelle Commissioni competenti, la 1a e la 2a, hanno ascoltato le audizioni rispetto alla alla condizione del Comune di Caivano e di Parco Verde. Molti del Gruppo cui appartengo, il MoVimento 5 Stelle, non paghi di ascoltare semplicemente attraverso il racconto come si vive in quei luoghi, hanno scelto di recarvisi perché non si può comprendere davvero come si vive e che Italia esiste al di sotto dell'Italia che si vede ad occhio nudo, ad occhio nudo, per poter guardare negli occhi le persone che vivono tutti i giorni in quella realtà. Abbiamo guardato negli occhi i dirigenti scolastici; abbiamo guardato negli occhi non solo don Patriciello, ma anche gli altri parroci che tanto fanno per quella comunità, i docenti e le Forze dell'ordine che in quel contesto devono lavorare. Presidente, le chiederei per favore di ottenere un po' di silenzio in Aula. PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di diminuire il tono della voce, come lo avevo chiesto prima, quando è intervenuto il senatore Gasparri, e non è stato fatto, senatrice. Quelle persone con cui abbiamo parlato non ci hanno rivolto delle richieste, ma delle preghiere. Ci hanno pregato di non dimenticarci di loro e non hanno fatto distinzione tra maggioranza e opposizione, Governo, Parlamento, perché per loro non significa nulla. Si sono rivolte alla politica, si sono rivolte a chi è nella posizione di poter fare qualcosa e ci hanno pregato di non dimenticarci di loro, quando il faro dei riflettori che adesso è acceso su Caivano, perché siamo in fase di conversione di questo decreto, si spegnerà. Il MoVimento 5 Stelle intende onorare la promessa che ha fatto: noi non ci dimenticheremo degli abitanti di Caivano, così come non ci dimenticheremo delle tante Caivano che esistono in Italia, delle tantissime periferie, del degrado che purtroppo affligge il nostro Paese da Nord a Sud. *(Applausi)*. Questo è un impegno che il MoVimento 5 Stelle prende in maniera ufficiale. Perché ci stiamo occupando di Caivano? Perché il mese scorso, a settembre, si è scoperchiato un vaso davvero putrido e maleodorante, si è scoperto di violenze inaudite che bambine di dieci e dodici anni subiscono, attenzione, da parte di chi?

e riprodotta poi sul *web*. Sono davvero cose agghiaccianti. Se si pensa ad un'infanzia distrutta, rubata, annullata, penso che questa sia l'immagine più eloquente che si stampa nella mente di chiunque. Prima ho sentito il sottosegretario Ostellari ringraziare le opposizioni. Bene, ne prendiamo atto, sono ringraziamenti dovuti. Immaginate, se questo è il quadro, in quale brutale violenza vivono tutti i giorni

per fargli venire in mente che forse intensificare la rete dei centri antiviolenza in quei posti avrebbe potuto dare una mano. Ma sono tante tante le dimenticanze del Governo, provocate

tante dimenticanze, sì, è vero. L'intenso lavoro delle opposizioni poi ci viene anche rinfacciato: il senatore Gasparri ha detto che abbiamo emendato troppo. Meno male che abbiamo emendato,

ha urlato mentre diceva che questi sono bambini. Dove hanno conosciuto il sesso in quel modo? Come è possibile che abbiano conosciuto il sesso in quel modo? Da noi adulti, dai siti pornografici fatti a uso e consumo degli adulti. Spegnete i siti pornografici, ci ha chiesto don Patriciello, fate sì che non siano più accessibili ai bambini, in alcun modo. Come ha risposto il Governo? Dimenticandosene. Anche in questo caso c'è voluto l'intervento delle opposizioni. E attenzione, perché perché noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo astenuti sull'emendamento che introduceva la possibilità che Agcom e il Garante della *privacy* valutassero le modalità con cui i siti pornografici si devono dotare di un sistema per cui possono certificare l'età di chi vi accede, ma poi non c'è alcuna sanzione. Un passetto avanti, allora, sì, ma il coraggio dove lo avete? Ascoltate don Patriciello soltanto quando vi pare. Dov'è il coraggio? Però, questo stesso decreto per Caivano si chiama contrasto alla povertà educativa, al disagio giovanile e alla criminalità giovanile. Attenzione: ieri, per la

guarda caso, "non ci azzecca" che cosa? L'emendamento del MoVimento 5 Stelle, che proponeva l'introduzione della figura dello psicologo negli istituti scolastici: quello l'avete reso improponibile, quello "non ci azzeccava".

per sventolare una bandiera. Noi però ci siamo impegnati a non abbandonare le persone di Caivano, le donne, le bambine, gli uomini e i ragazzi

allora, che noi la fiducia a questo Governo non la possiamo dare e che diciamo no alla vostra arroganza, no al vostro militarismo e no a voi che gli ultimi li avete abbandonati,

Ci saremmo astenuti su questo provvedimento, però, signor Presidente, perché anche solo un briciolo di speranza che hanno gli abitanti di Caivano noi non la vogliamo spegnere, vigileremo: vigileremo ogni giorno che le vostre promesse non siano state

diffuse via cellulare; una giovane di diciassette anni si è suicidata, dopo essere stata vittima di violenza; una ragazza è stata stuprata la notte di capodanno e ha poi tentato di uccidersi; una tredicenne è stata aggredita con una forbice da due coetanei. Ecco, questi sono alcuni casi di cronaca

abbiamo preso ad esempio, quindi Caivano, ma anche distretti come quelli della stessa Milano. Il tema è delicatissimo e riguarda veramente i ragazzi, il loro comportamento e la difficoltà di affrontare il superamento dei limiti.

La situazione deve essere affrontata in maniera sinergica, lavorando insieme, facendo rete fra le Forze dell'ordine, i magistrati, gli operatori sociali, i gestori degli esercizi pubblici, la scuola, gli psicologi, i medici, gli amministratori, le associazioni.

l'innalzamento delle pene da diciotto mesi a cinque anni anche per spaccio di lieve entità, purché non occasionale; prevede un divieto, per chi usufruisce della sospensione condizionale in caso di spaccio in luoghi pubblici, di avere accesso proprio a quegli spazi pubblici, come le scuole.

sta già sbagliando. Ottima poi la misura (che avevamo già previsto nel nostro disegno di legge) della rieducazione del minore, in una fase che arriva prima dell'apertura del processo, prima della condanna, prima del carcere.

signori, non possiamo spaventarci di fronte a un ampliamento dell'applicazione dell'istituto della custodia cautelare. Stiamo parlando di reati quali l'omicidio e la rapina aggravata, non stiamo parlando del furto di una mela.

è fra l'esecuzione della pena e la rieducazione, non la contrapposizione galera sì, galera no. Non poniamo le questioni in maniera semplicistica. Il fenomeno della delinquenza minorile, come ha detto, appunto, il sottosegretario Ostellari, non è scoppiato sei mesi fa. Questi sono i dati che noi abbiamo. Se ci sono quasi 450 detenuti minori in carcere, si vede che qualcosa è successo prima e che nessuno ha fatto I binari sui quali costruire un sistema sono binari che si inseriscono su un percorso: l'ammonimento, l'avviso orale, il Daspo, la lotta contro l'abbandono scolastico. Questi sono solo degli elementi che si inseriscono su un processo minorile che va riformato, e questi sono alcuni dei passi per riformarlo.

sono stati fatti degli interventi anche per recuperare queste strutture carcerarie. Riconosciamo che questo Governo ha finalmente messo mano a una problematica, cioè le strutture carcerarie, carcerarie, ma non per creare meri istituti penitenziari, bensì nuove strutture, più vicine al concetto della comunità, per fare rieducazione, se non addirittura educazione. Questa è una delle risposte, quella relativa alle strutture, e altre risposte sono contenute all'interno di questo decreto. Non esiste, però, una soluzione unica, valida per tutti. Con la liberalizzazione della droga non risolviamo il problema della droga fra i giovani,

Occorre fare delle analisi serie, guardandoci veramente in faccia. Forse questo provvedimento non è quello che risolverà tutte le problematiche giovanili, ma è una risposta importante e decisa, che noi condividiamo. Per questa ragione, tutto il Gruppo della Lega voterà convintamente la fiducia.

Intanto, vorrei iniziare sgomberando subito il campo da qualche ambiguità e da qualche dubbio. Noi consideriamo la vicenda di Caivano, quel contesto così tragicamente descritto dagli episodi di cronaca e anche dalle testimonianze, che abbiamo ascoltato in Commissione, di don Patriciello, come un contesto che ci obbliga a fare i conti con le condizioni di disagio, di delinquenza e di criminalità che affliggono, non solo Caivano, ma tante periferie del nostro Paese. Non c'è dubbio, lo ammettiamo, che il disagio giovanile, che effettivamente è cresciuto moltissimo, soprattutto dopo la pandemia, le sue proiezioni sul piano delle condotte illecite, che sono aumentate in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni, creino allarme nell'opinione pubblica e che devono essere al centro delle nostre preoccupazioni, anche come legislatori. Proprio per questo, cari colleghi, proprio perché ci troviamo a trattare e occuparci di un tema così delicato, riguardante i minori, i nostri ragazzi e il futuro del nostro Paese, non si fa così. Non si fa con un decreto-legge. Non si fa con uno strumento che impedisce una discussione. *(Applausi)*. Abbiamo visto come abbiamo dovuto lavorare, caro Presidente della 1ª Commissione. In un giorno abbiamo dovuto svolgere quindici audizioni per riuscire a stare nei tempi. Abbiamo fatto le corse in Commissione. Ieri c'è stata una confusione drammatica sulle riformulazioni degli emendamenti e sui pareri agli emendamenti. Abbiamo aspettato due ore in Commissione che il Governo decidesse qualcosa su un emendamento improvvisamente comparso, che non c'entra nulla con il decreto Caivano e che riguarda le società di calcio della serie A e la pirateria informatica. Vi abbiamo garantito i tempi per arrivare in Aula: altro che ostruzionismo, senatore Gasparri. *(Applausi)*. È meglio tacere, invece di insultare l'opposizione, se non si conosce il contenuto del provvedimento e come ci si è arrivati. Non abbiamo fatto alcun ostruzionismo e ce ne dovete dare atto. È umiliante per tutti, per noi dell'opposizione ma anche per voi della maggioranza, dover lavorare in questo modo. Non si possono sacrificare sempre il confronto, l'approfondimento, la cura nella scelta e nella redazione di norme che toccano la carne viva delle persone; non si può sacrificare tutto questo sull'altare del messaggio mediatico, del segnale da mandare all'opinione pubblica, del solito vizio nel quale incorrete, incuranti degli effetti delle vostre scelte. Questo è il punto: come come si combatte davvero il disagio e la criminalità minorile; come si aiutano i ragazzi a uscire da una spirale di degrado che li porta sulla strada della criminalità. Ci sono due versanti della risposta, che però si tengono: uno è la repressione, che però - attenzione - deve essere strettamente finalizzata all'assunzione di responsabilità da parte del minore e al suo recupero; riguarda tutto l'apparato di interventi di natura preventiva, orientati alla cura dei profili educativi dei ragazzi e a un ampliamento delle politiche sociali. Voi avete scelto la repressione e vi siete dimenticati di tutto il resto. Il nostro diritto penale minorile è un fiore all'occhiello della giustizia italiana, proprio per gli istituti e le misure volte al recupero del minore,

Ebbene, cosa avete fatto? Lo ricordo al Sottosegretario, che oggi se n'è dimenticato, quando ha fatto il suo intervento in replica. Avete aumentato a dismisura la possibilità di applicare ai minori le misure cautelari, compresa la custodia cautelare, e la loro durata; avete aumentato le pene per diversi reati; avete allargato ai minori le misure di sicurezza urbana che si applicavano ai maggiorenni; con gli emendamenti in sede di istruttoria siete addirittura riusciti a peggiorare il testo, riducendo il perimetro di applicazione dello strumento più efficace per recuperare i minori, ossia la messa alla prova; avete reso addirittura più facile l'ingresso in carcere per i minori che creano problemi nelle case di comunità. La vostra risposta è la solita anche per i minori: più carcere. *(Applausi)*. Come ci hanno detto le camere penali, siete riusciti a trascinare anche il sistema della giustizia minorile, finora risparmiata da interventi demagogici e disorganici, verso una deriva panpenalistica e carcerocentrica. Il garante uscente dei detenuti Mauro Palma, al quale abbiamo al quale abbiamo chiesto che impatto avranno queste misure sui penitenziari minorili, ci ha detto che queste misure comporteranno un aumento dei detenuti negli istituti penitenziari minorili del 20 per in strutture già al limite della capienza. Dunque vi chiedo - non c'è il Sottosegretario, altrimenti chiederei a lui - cosa c'è in questo decreto-legge per migliorare gli istituti penitenziari minorili per incrementare le case di comunità, per rendere più efficace e capillare la messa alla prova e gli altri istituti volti alla responsabilizzazione e al recupero del minore. Cosa c'è in questo decreto? Zero *(Applausi)*, non c'è niente, niente di niente. Li buttate in carcere e lì finisce il vostro intervento. Pensate che questa sia la soluzione? Non capite che con più ragazzi in carcere, senza alcuna prospettiva, aumenta solo il rischio di consegnarli per sempre alla deriva criminale? Come ci ha detto la presidente dei magistrati minorili italiani, questi interventi, lungi dal risolvere il problema - che c'è - del disagio e della criminalità minorile, rischiano solo di aprire crepe irreversibili in un sistema che tutta l'Europa ci invidia. allora provato a lavorare su un altro versante e abbiamo provato a capire se almeno sotto il fronte degli interventi di prevenzione, di presenza di presidi educativi, di biblioteche di territorio, di presa in carico delle famiglie disagiate, di aumento dei servizi sociali e di comunità, ci fosse la possibilità di intervenire. Abbiamo presentato decine di emendamenti, ma ci avete risposto

per la videosorveglianza. Vi pare possibile intervenire in questo modo? Perfino gli emendamenti dei relatori, che cercavano timidamente di far piccoli passi in avanti su questo terreno, sono stati precipitosamente ritirati per mancanza di disponibilità. Non ci sono risorse per la prevenzione, non ci sono risorse per l'educazione, non ci sono risorse per le case di comunità, non ci sono risorse per le misure alternative alla detenzione. In buona sostanza, non c'è nulla di quello che serve. *(Applausi)*. Non contenti, Non contenti, avete anche deciso di cogliere l'occasione per aumentare le pene per il reato di traffico di stupefacenti di lieve entità. Chi vi parla non è un sostenitore della liberalizzazione e della depenalizzazione: qui però voi avete fatto una cosa che produrrà degli effetti, perché avete aumentato la pena per quei reati di lieve entità da quattro a cinque anni e questo comporterà l'arresto obbligatorio in flagranza e la custodia cautelare, con il rischio di un impatto sulla popolazione carceraria di diverse migliaia di unità. Noi abbiamo chiesto ripetutamente al Sottosegretario di avere una stima dell'impatto che avrà questa misura, ma non ci ha risposto. Il rischio è quello, perché noi sappiamo che quando è stata diminuita quella pena negli anni passati, ciò ha consentito di deflazionare la popolazione carceraria. Ora, se l'effetto sarà quello, non venite poi a versare lacrime di coccodrillo quando ci saranno episodi drammatici nelle carceri italiane dovuti al sovraffollamento *(Applausi)*, perché sappiamo di chi sarà la colpa. conclusione, Presidente, noi siamo molto rammaricati per il metodo e le modalità consuete con le quali si è intervenuti. È un'occasione perduta e siamo anche fortemente preoccupati per questi interventi che rischiano di scardinare il nostro sistema penale minorile.

Voglio chiudere con le parole di Don Ciotti a proposito dei ragazzi, del loro disagio e dei contesti di degrado in cui spesso vivono: «L'esercito di cui hanno bisogno lì deve essere composto da educatori, assistenti sociali, operatori della cultura. Bisogna costruire opportunità, fornire strumenti e servizi. Questa è l'unica via d'uscita». Di tutto questo, in questo decreto-legge, non c'è traccia e per questo voteremo contro.

pone all'Aula una grande responsabilità, in primo luogo perché il Governo vi ha posto la questione di fiducia e quindi, secondo la prassi costituzionale e le regole parlamentari, ritiene questo provvedimento fondamentale e alla sua approvazione subordina la sua stessa permanenza in carica. *(Applausi)* Pone poi responsabilità per questioni di stretto merito, per la filosofia che lo ispira, per la complessità della materia, per le ragioni che lo giustificano e anche e soprattutto per i destinatari delle sue disposizioni, che sono da un lato la tutela e la sopravvivenza delle nostre periferie, dall'altro il futuro dei nostri minorenni. Perché questo - badate - è un provvedimento di contrasto, ma di contrasto in primo luogo al disagio e al degrado sociale, alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e allo stesso diviene strumento di contrasto durissimo alla devianza e alla criminalità minorile, che hanno assunto in Italia un grado di pervicacia che ha determinato un enorme allarme sociale. Ebbene, dinanzi a questo scenario e a questa responsabilità, ci si attende che ai pensieri, sempre nobili, soprattutto qui in quest'Aula sovrana, non debbano seguire solo parole, ma anche fatti. Invece, ad ascoltare le dichiarazioni di voto delle opposizioni, sembra - per dirla con Schopenhauer che i pensieri comincino a morire nel momento stesso in cui prendono forma le parole. *(Applausi)*. Dalle vostre parole, infatti, si intende perfettamente che non avete compreso cosa sta accadendo nelle tante Caivano d'Italia Nessuno dalle opposizioni ha compreso quale degrado imperante stia avvolgendo le nostre periferie. Nessuno dalle opposizioni ha compreso che a Caivano, come nelle tante Caivano d'Italia, si sta registrando il fallimento della politica, il collasso culturale, la resa delle istituzioni ed è una circostanza che non ci possiamo più permettere. Molti di voi probabilmente non sono mai stati a Caivano e non ci andranno mai, magari non sanno neppure dove sia, ma in quel luogo di 35.000 anime è accaduto l'inverosimile, quel luogo è divenuto la piazza di spaccio più grande d'Europa, un luogo presidiato soltanto dalle vedette della camorra, un luogo - per dirlo con le parole di don Patriciello - in cui per attraversare il centro del paese bisogna percorrere cinque piazze di spaccio diverse ed è intollerabile che fino a ieri, fino ai nostri interventi, a presidiare le istituzioni siano rimasti soltanto un piccolo, coraggioso parroco di provincia ed un capitano dei Carabinieri. E questo è accaduto nel silenzio della politica, perché in quella terra martoriata noi abbiamo un'amministrazione regionale silente e quindi complice, un'amministrazione metropolitana catatonica e quindi inutile, abbiamo un'amministrazione comunale infiltrata e pertanto letale. *(Applausi)*. È inevitabile, allora, che Caivano sia divenuta un concentrato di omertà, illegalità, degrado, infanzia violata. A fronte di questo scenario e di questa responsabilità, non possiamo più permetterci filosofie teoretiche, giustificazionismi sociali e pelosi o sociologia di accatto *(Applausi)*. Noi dobbiamo assumere provvedimenti, dobbiamo fare in modo che seguano i fatti ed il provvedimento in conversione va esattamente in questa direzione.

e non bisogna aver paura di aver coraggio, al contrario bisogna agire con il cuore al fianco di intere comunità ferite ed oltraggiate. *(Applausi)*. È un provvedimento e *libra* - bilancia - uguali sulla bilancia) perché riesce a coniugare e a bilanciare prevenzione e repressione, legalità e socialità, rigore e garanzie, rispetto e merito,

lo Stato non si può permettere di arretrare neppure di un passo. *(Applausi)*. E vi dico di più e lo dico da napoletano innamorato della propria terra, eletto in quella valle di lacrime: è un provvedimento del quale siamo grati al Governo e al Presidente del Consiglio. *(Applausi)*. È un provvedimento del quale siamo fieri dinanzi all'Italia perché cambia il paradigma, permettendo finalmente di approntare una risposta reale a territori abbandonati e di contrastare duramente la criminalità minorile, ferma restando la specificità del minore e quindi immaginando percorsi di accompagnamento e di recupero, senza però cedimento alcuno nei confronti di chi delinque. I provvedimenti vanno tutti in questa direzione; non sono misure penali, sono misure che anticipano la soglia penale, che vogliono agire sul fronte della prevenzione. Come? Attraverso tutti gli articoli che lo disciplinano, aumentando il livello di sicurezza pubblica, rafforzando la tutela dei centri urbani, ampliando misure straordinarie che restituiscono alle amministrazioni locali, alla polizia di sicurezza ai sindaci del territorio una serie di strumenti formidabili per anticipare la soglia della tutela penale ed intervenire prima che la devianza diventi criminalità. ampliamento del foglio di via obbligatorio; fuori da quei territori chi non è degno di starci *(Applausi)*, ammonimento orale, avviso del questore, misure di prevenzione anche per i minorenni perché non è più tollerabile quella deriva. È tutta una serie di misure accessorie che vanno a stringere il campo dello spaccio di stupefacenti, restringendo la possibilità di muoversi liberamente con le armi su quel territorio ed incidendo su un reato odioso e vigliacco che è quello della stesa *(Applausi)* attraverso cui criminali in armi tengono in ostaggio intere comunità che aspettano soltanto di essere affrancate. se fosse tutto qui, ci sarebbe soltanto il fronte della repressione o della precautela, ma il decreto-legge interviene con molti articoli sul fronte complementare. È un provvedimento a doppia matrice,

ed investire fortemente con degli stanziamenti sulla dispersione scolastica, punire e sanzionare chi, in veste della propria figura di custode e di responsabile genitoriale, abbandona i ragazzi al loro destino. stanzia dei fondi complementari a quelli dell'Agenda Sud per avere una speranza di riscatto. Se questo è lo scenario, noi siamo consapevoli che solo la responsabilizzazione pone il Paese dinanzi a una prospettiva di benessere sociale. Il minore che delinque però interiorizzare la cultura del rispetto, deve comprendere fino in fondo che il reato, se commesso, deve diventare l'occasione per un ripensamento stesso della propria condotta e del disvalore sociale e morale delle proprie azioni. Soltanto attraverso la cura e l'esercizio dei diritti sarà possibile coniugare il puntuale adempimento dei doveri. Signori, per noi questa è l'unica strada possibile. Le avete percorse tutte, tutte fallimentari; è l'unica strada che ci resta per recuperare territori e comunità allo Stato *(Applausi)*, per chiudere con le zone franche, per recuperare e tutelare i nostri minori. È l'unica strada possibile. È vero, Caivano è una disperazione, bisogna a volte attraversare i sentieri della notte per vedere l'alba. Ebbene l'alba è prossima, l'alba è giunta e noi la salutiamo con il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(È estratto a

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023,

Presidente, intervengo per portare a conoscenza dell'Aula che dal 18 ottobre 2023, dopo una conferenza stampa presso la Camera dei deputati del Movimento degli allevatori meridionale, in cui si annunciava l'inizio di uno sciopero della fame per sostenere la richiesta della nomina di un Commissario nazionale sulla brucellosi e la TBC nelle Regioni meridionali, in due Regioni, Campania e Sicilia, lo sciopero è in corso: Pasquale D'Agostino in Campania e Sebastiano Lombardo in Sicilia sono al loro nono giorno di sciopero della fame e hanno annunciato che non si fermeranno fino a quando il Governo nazionale non avrà dato una risposta. Si chiede al Governo di intervenire, indicando le direttrici su cui riorganizzare e risolvere problemi che da decenni stanno tenendo le aree rurali e il comparto produttivo allevatoriale nella crisi. I numeri, mai smentiti, sono diventati consapevolezza dell'opinione pubblica nazionale, dopo che sono emersi grazie a inchieste giornalistiche e all'azione continua degli allevatori di bufala casertani ed ora, grazie all'indagine conoscitiva